Signor Presidente, onorevoli colleghi, la grave crisi che ha investito in questi ultimi mesi i mercati finanziari ha reso necessario l'intervento di tutti i Governi internazionali per arginare le perdite accumulate dagli istituti di credito.

Il Governo del nostro Paese ha predisposto un disegno di legge che amo definire salva banche.

quelli che servono al Paese, che non è di destra né di sinistra. Il nostro è un Paese che sta aspettando ancora le riforme necessarie per decollare,

Il decreto che siamo chiamati a convertire, che serve per ricapitalizzare le banche in crisi, è nato tra mille dubbi,

esiste la necessità di decidere come, quando, dove e perché dobbiamo incontrarci, perché insieme dobbiamo tentare di dare una soluzione reale ai problemi della nostra terra che è una ed è inscindibile,

alle famiglie con le tessere di povertà di antica memoria sono una cosa giusta e sacrosanta, che hanno un aspetto positivo.

se vogliamo trovare un punto di incontro serio non c'è bisogno di fare un tavolo con un sindacato in casa ad Arcore e un altro con un altro sindacato in altra sede. C'è la necessità di incontrarci qua, nelle Commissioni o in Aula, per stabilire un contatto diverso tra maggioranza e minoranza e tentare tutti insieme di compiere un dovere sacrosanto, che è quello di ridare credibilità alle istituzioni e assicurare a chi soffre

signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, avevamo presentato alcuni significativi emendamenti al vostro decreto cosiddetto con la finalità di migliorarne gli effetti ed offrire alcune tangibili garanzie alle famiglie ed alle piccole e medie imprese che soffrono i morsi della crisi; ma questi non sono stati accolti salvo la trasformazione, per alcuni, in ordini del giorno che - come è noto - non hanno alcun effetto reale. Avevamo chiesto negli emendamenti di abrogare l'istituto della commissione di massimo scoperto, un vero e proprio «pizzo» che aggrava il costo del credito, secondo Bankitalia del 4,37 per cento su base annua (ossia anche del 43 per cento su un affidamento regolato al 10 per cento) costringendo le piccole e medie imprese ma anche lavoratori e pensionati poco attenti al gioco delle valute, a corrispondere decine, a volte centinaia se non migliaia di euro su assegni scoperti di valuta anche per un solo giorno. Avevamo chiesto di sostenere tre milioni e duecentomila famiglie indebitate a tasso variabile per precise responsabilità delle banche, quando i tassi BCE nel 2004 e 2005 erano al 2 per cento e tutti gli indicatori economici propendevano per un loro imminente aumento. Avevamo chiesto di mettere argine allo strapotere di istituti di credito che non si fidano di se stessi ed hanno la pretesa che consumatori ed imprese possano fidarsi di loro, che utilizza le centinaia di miliardi di liquidità provenienti dalla BCE non nel mercato interbancario, ma nei conti *overnight* aperti dalla stessa Banca centrale, chiedendo invece la revoca dell'affidamento ed il rientro dei fidi con un preavviso di 24 ore. Avevamo chiesto che l'oro e le riserve di Bankitalia fossero dismesse per contribuire al risanamento ed alla riduzione del debito pubblico, così come hanno fatto tutti i Paesi dell'area euro, e che le quote di partecipazione delle banche in Bankitalia, che determinano un enorme conflitto di interesse tra vigilanti e vigilati, fossero rimborsate al valore nominale maggiorato e rivalutato secondo gli indici ISTAT. Avevamo chiesto che anche ai membri del consiglio di amministrazione delle banche, per i quali il Governo vara un salvacondotto di garanzia per le loro malefatte a danno - lo ripeto - di un milione di risparmiatori ai quali sono stati appioppati polizze tossiche e *bond* bidone già all'origine avariati (da Cirio a Parmalat, da quelli argentini a Lehman Brothers), quindi agli esecutivi ed ai dirigenti apicali fossero ridotti del 10 per cento i loro ricchi emolumenti. Ricordo ancora di banchieri anno hanno guadagnato 26-27.000 euro al giorno, oltre a 450.000 azioni della propria banca. Avevamo chiesto che vi fossero garanzie per quei risparmiatori i quali, fidandosi dei cattivi consigli delle banche, hanno investito il loro sudato risparmio nel paniere di titoli promosso da Patti chiari, il consorzio dell'ABI (Associazione bancaria

Avevamo chiesto l'istituzione di una commissione bicamerale di vigilanza sulla stabilità del sistema bancario ed una data certa per l'attivazione della *class action*, formidabile strumento di deterrenza contro i tanti furbetti del quartierino, nonché regolatrice del mercato per chi crede alla concorrenza. Il decreto salva banche - mi dispiace dirlo - non ha recepito nulla di tutto questo, con la giustificazione che alcuni di questi emendamenti, certo incentivi per chi piazza *bond* bidone, ma affidamenti di qualità alle piccole e medie imprese, seppur giusti e condivisi, sono prematuri e forse accoglibili in un futuro che non arriverà mai. Signori rappresentanti del Governo, se questo vostro decreto doveva servire ad arginare le turbolenze dei mercati, basta vedere gli andamenti di borsa per avere risposte. Se doveva servire a restituire la fiducia tradita, segnalo che mentre la BCE taglia il costo del denaro, colossi primari devono aumentare i rendimenti per piazzare alcuni *bond*, perché o restano invenduti (quelli di primarie banche) oppure, per essere collocati, devono garantire altissimi rendimenti. L'ENI, che è un colosso, per collocare la sua ultima emissione di 1,25 miliardi, ha dovuto offrire un rendimento molto elevato,

E per le banche italiane che hanno emesso montagne di *bond*, pari, al 30 settembre, alla cifra record di 718 miliardi di euro, ossia 2,6 volte patrimonio e riserve, non sarà facile rinnovare tali scadenze. Ricordo, infatti, che le obbligazioni bancarie, voce negativa del bilancio patrimoniale, ossia debiti rappresentati da titoli con scadenze e rendimenti, corrispondono quasi al triplo del capitale e delle riserve. Nei prossimi 14 mesi circa un quinto di questo gigantesco monte di obbligazioni, ossia 135,5 miliardi di euro, andrà in scadenza: entro dicembre 2008 e 110,4 miliardi nel 2009. Secondo i dati di Bloomberg, tra ottobre 2008 e dicembre 2009 *bond* per 42 miliardi andranno in scadenza per Unicredit; 32 per Bancaintesa; 20 per Monpaschi, 15 miliardi per UBI Banca; 11,4 per il Banco Popolare; 6,2 per Bnl-Paribas; 5 per Mediobanca; 3,6 per Banca popolare di Milano. Nel 2010 matureranno ulteriori *bond* per 100 miliardi di euro, dei quali 36 per Unicredit e 31 per Intesa, mentre entro il 2013 gli otto maggiori gruppi bancari, Unicredit, Intesa, Monpaschi, Ubi, Banco popolare, Bnl, Mediobanca e Bpm, dovranno rifinanziare obbligazioni proprie per 429 miliardi. Signora Presidente, onorevoli colleghi, per queste ragioni,

che andavano verso una maggiore trasparenza e garanzia dei diritti dei consumatori e dei risparmiatori. Ci dispiace, signora Presidente, signora Presidente, signori del Governo, di non poter votare un provvedimento che salva le banche, offre un salvacondotto ai banchieri e ai bancarottieri, ma affossa le famiglie e le piccole e medie imprese che avevano bisogno di un aiuto tangibile per potersi risollevare, oltre la carta di carità. *(Applausi Signora Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, la crisi finanziaria che sta devastando i mercati dei capitali era iniziata nell'agosto del 2007 come crisi del mercato dei mutui *subprime*; si è sviluppata in seguito come crisi di un modello di intermediazione, quello delle banche di investimento di Wall Street; infine dal mese di settembre è deflagrata come una vera e propria crisi bancaria investendo anche l'Europa e i sistemi finanziari dei mercati emergenti. Possiamo individuare tre cause principali: sicuramente un allentamento delle regole dell'intermediazione, basato sulla convinzione che una volta assicurata la stabilità del sistema bancario e protetti i depositanti al dettaglio, il sistema finanziario non avesse bisogno di altre regole e potesse fare da sé; poi un crescente deterioramento degli standard di credito, soprattutto, ma non solo, per i mutui immobiliari, in larga parte guidato dalle due grandi agenzie parapubbliche di mutui immobiliari, Fannie Mae e Freddie Mac; infine, la creazione di una fabbrica di alti rendimenti in un contesto di bassi tassi d'interesse. Di fronte a questa deflagrazione, il Governo ha saputo intervenire con prontezza e decisione con il provvedimento che ora è all'approvazione da parte del Parlamento, secondo un modello di garanzia, di sicurezza e di stabilità del sistema creditizio; non mi piace chiamare questo decreto legislativo salva banche, ma Per quanto riguarda la sicurezza, direi proprio che questo è il *know-how* che la Lega ha portato e porta come valore aggiunto all'interno del Governo e della coalizione che governa, il Paese. Con questo decreto, dunque, si vuole aumentare la stabilità del sistema del credito, incrementare le contrattazioni nel mercato dei prestiti interbancari e soprattutto, cosa non da poco, favorire la solvibilità delle banche per garantire il flusso dell'economia reale, questo è il nodo fondamentale per lo sviluppo: riportare l'attenzione sull'economia reale, non su un'economia virtuale e di tipo finanziario. Il punto è proprio questo: l'economia reale, che è già influenzata negativamente dalla bufera infuriata in questi giorni nelle borse mondiali, deve essere assolutamente tutelata e salvaguardata. La domanda è: chi può farlo se non il nostro Governo, che si sta muovendo con attenzione nei confronti del mondo reale mondo reale che potrei definire, visto che parliamo di questioni di tipo finanziario, il *core business* politico della Lega, che sono appunto le famiglie, i lavoratori, le piccole e medie imprese; è il cittadino, è la nostra comunità, la nostra collettività. Noi siamo in questo Governo, in questo Parlamento, nella maggioranza per garantire questi nostri punti di riferimento per il Nord e per tutto il Paese. Ringraziamo anche

Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, anche in questo caso siamo chiamati in «zona Cesarini» a convertire un provvedimento, su cui, come Senato, abbiamo avuto pochissimo spazio per discussione e confronto. Ci è stato risposto che questo potrà avvenire meglio su altri provvedimenti, come il decreto-legge n. 185, vedremo! Certo è un po' singolare che non sia mai il momento per una vera disamina del merito, che ogni volta si rinvii alla scadenza che verrà.

dalla necessità di far fronte agli sconvolgimenti derivanti dalla crisi finanziaria in atto, adottando misure tese a garantire la stabilità del sistema bancario e, per questa via, ad assicurare la tutela del risparmio, così duramente colpito e penalizzato. Ci sarà più tempo e spazio, quando discuteremo la mozione presentata dal nostro come da altri Gruppi, per analizzare le ragioni che hanno portato a questa gravissima crisi, che non è solo finanziaria, ma è fondamentalmente economica, come ha ben spiegato ieri, nel suo intervento, il senatore Morando. Qui valga semplicemente sottolineare che le sue cause profonde stanno in quei due drammatici squilibri: la gravissima carenza di risparmio negli Stati Uniti e la forte eccedenza di risparmio nelle economie emergenti. Certo, come è risultato evidente Certo, come è risultato evidente anche dall'indagine condotta dalla nostra Commissione sulla materia, alla base di questa crisi ci sono altresì specifiche scelte delle istituzioni politiche e delle autorità dì regolazione. Si è colpevolmente lasciato crescere un sistema finanziario quasi parallelo, in cui le banche più grandi e più sofisticate hanno potuto spogliarsi di una gran parte del rischio di credito, ingenerando una vera e propria illusione che per il rischio, i vincoli di bilancio e la scarsità di risorse ci fosse sempre un altro stadio cui trasferirli. Quando, a furia di frullare, la maionese è impazzita, l'inganno si è svelato e i mercati sono rimasti nudi. Oggi regna l'instabilità, l'incertezza, la sfiducia, ma, soprattutto, gli effetti della crisi finanziaria in atto si stanno trasferendo nell'economia globale e investono direttamente l'Europa, dove pure il dissolversi della fiducia nei mercati può causare, e sta causando, gravi danni all'economia reale, minacciando posti di lavoro e la sopravvivenza di molte imprese. La natura del provvedimento di cui ci occupiamo si iscrive in questo quadro: fornire opportunamente una rassicurazione ai risparmiatori; dare stabilità al sistema del credito; attrezzarsi nel caso di evenienze particolarmente negative di singole aziende bancarie. Tuttavia, questo provvedimento, che nella logica che lo ha motivato possiamo condividere e che abbiamo, nella discussione più di merito svoltasi alla Camera, contribuito a migliorare (avremmo voluto farlo anche qui, ma non ce n'è stata la possibilità), ha ormai esaurito - come ha ammesso anche il rappresentante del Governo - la sua spinta propulsiva, che è stata sostanzialmente una funzione di rassicurazione e stabilizzazione, senza grandi implicazioni di carattere operativo, a conferma che i processi evolvono con una rapidità straordinaria e che la tempestività è una condizione del risultato che si può provare a conseguire. In questo senso, dissentiamo, e grandemente, per quel che non c'è nel decreto. se le misure del Governo appaiono sufficientemente appropriate a conseguire gli obiettivi sul fronte della tutela del risparmio, altrettanto non può dirsi per l'esigenza di assicurare continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, alla luce anche delle analisi recentemente condotte dalla Banca d'Italia sul persistere di una generale crisi di liquidità del nostro sistema. c'è la necessità, specie dopo il dissesto della banca d'affari Lehman Brothers, vero spartiacque nel precipitare della crisi su scala generale, di ricostruire la fluidità del circuito interbancario, ma nel contesto delle criticità europee c'è una specificità tutta italiana. Paradossalmente, anche *asset* più positivi che noi potremmo avere stanno giocando in negativo, perché gli istituti bancari del nostro Paese, dato che stanno un po' meglio dei loro competitori europei, non hanno dovuto o voluto o comunque si sono astenuti dal far ricorso all'intervento di ultima istanza dello Stato, né tanto meno hanno acceduto agli strumenti forniti col decreto che oggi è all'attenzione dell'Aula. stanno così cercando di migliorare i loro coefficienti patrimoniali (operazione che comunque è indispensabile fare) restringendo il credito. Ciò fa sì che la tendenza recessiva in Italia si è innescata e sta procedendo molto più velocemente e automaticamente di quanto non sia avvenuto o stia avvenendo in altri Paesi europei. Insomma, siamo meno coinvolti nella crisi finanziaria, ma, per le nostre debolezze strutturali e non solo, le ricadute di questa sull'economia reale procedono più velocemente. Anche per questo, signor rappresentante del Governo, occorre mettere in campo misure che incidano e invertano o almeno frenino la situazione. Chissà se anche nel Governo qualcuno ha cominciato a pentirsi per aver, in questi mesi, sostanzialmente dissipato risorse con scelte discutibili e miopi: dai due dai due miliardi e mezzo di soppressione dell'ICI sulla prima casa per i ceti abbienti, al costo dell'operazione di salvataggio dell'Alitalia, dopo aver lasciato per strada soluzioni molto più a buon mercato, al drastico abbassamento dell'asticella della fedeltà fiscale (a partire da quella tracciabilità dei pagamenti, di cui stamattina per fortuna abbiamo visto un piccolo segno di resipiscenza). Il tema di oggi non è solo quello della crisi finanziaria; occorre affrontare la questione del sostegno all'economia reale e di come procedere con misure anti-recessive. In questo senso, come Partito Democratico, noi insistiamo perché sulle risorse che il Governo destina o potrebbe impiegare a favore del sistema creditizio si eserciti uno scrupoloso controllo

possano trattare meglio nei rapporti con gli istituti bancari, investendo e rafforzando il ruolo dei confidi. Ma perché le misure siano efficaci bisogna metterci fondi, soldi veri, non limitarsi alla *moral suasion*. Ci vogliono interventi strutturali, e non *una tantum*, su salari, pensioni e stipendi medio-bassi. Faccio notare che quest'anno la percentuale di entrate da tassazione del lavoro dipendente e delle pensioni toccherà il livello record sul totale del gettito. Come pensate che si possano rilanciare i consumi senza un intervento serio, non elemosine, in questa direzione? Ci vuole, infine, un piano credibile di investimenti pubblici, e perché almeno una parte sia accantierabile subito, se vi fidate dell'esperienza di chi un po' di amministrazione l'ha praticata, ci vuole l'intervento di Enti locali e Regioni, gli unici in grado di garantirlo, rimuovendo alcune rigidità del patto di stabilità come stiamo chiedendo nella discussione sulla finanziaria. Ma voi vi muovete su un altro registro. Tra le misure disposte col decreto-legge n. 185, di cui discuteremo, ce n'è una davvero emblematica. Mi riferisco alle norma che riduce la detraibilità del 55 per cento per gli interventi per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale. Mi pare davvero una perla di insipienza, se posso permettermi; si colpisce una misura utile, che fa risparmiare energia e costi, che può innescare un volano per tante piccole e medie imprese: a che pro? Andrebbe incentivata e invece si perpetra uno scippo e consistente a danno di tanti cittadini, cambiando le carte in tavola. Si restringe e si burocratizza, alla faccia della semplificazione. E con lo Statuto del contribuente e il vincolo a non adottare norme con valore retroattivo come la mettiamo in caso? Mi ricordo in quest'Aula, nei due anni precedenti, le intemerate nei confronti del fisco vampiro del Governo Prodi e Visco e mi ricordo le lezioni su come creare convergenze di interessi

vuole che si comunichi fiducia agli italiani, forse dovrebbe tenere un po' più a bada il suo Ministro, perché questi interventi segnano a fondo la fiducia dei cittadini. Noi, come Partito Noi, come Partito Democratico, ci asteniamo dal voto del provvedimento, perchè vogliamo così rimarcare quel che in esso non c'è, evidenziare i vostri ritardi e le vostre responsabilità, incalzarvi per un cambio di indirizzo nella politica economica nell'interesse del Paese.

onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo PdL vorrei svolgere tre rapidissime La prima riguarda le motivazioni con cui alcuni Gruppi hanno espresso la loro contrarietà, che si esprimerà in un voto di astensione nel merito del provvedimento,

collega Cintola. Tutti i rappresentanti qui presenti del Gruppo del Popolo della Libertà non sono automi che spingono i bottoni e fanno accendere le lucette: sono cittadini italiani eletti dal popolo e responsabili del loro comportamento. Quindi, la prego, senatore Cintola, di non usare più questi riferimenti ad automi automatici.

Quindi, l'effetto vero di questo decreto è sotto gli occhi di tutti, cioè quello che non è accaduto in quei giorni. Questo decreto ha svolto positivamente ed egregiamente il suo ruolo ed il suo compito, che era quello non di salvare le banche, ma di dare assicurazioni ai depositanti ed ai risparmiatori per evitare il panico. *(Applausi dal Gruppo PdL).* Altro che salva banche: salva famiglie, salva imprese, salva depositanti; e questo effetto si è già realizzato, cari colleghi dell'opposizione o del Senato in genere:

che la crisi finanziaria si avviti nella crisi dell'economia reale. Ebbene, se così è,

È sotto gli occhi di tutti che il rischio che ci sia una restrizione creditizia è totalmente legato al blocco del mercato interbancario e sul mercato interbancario è urgente che la Banca centrale europea, oltre ad abbassare efficacemente i tassi di interesse, conceda garanzie affinché le banche tornino a fidarsi tra loro, altrimenti tutti i provvedimenti suggeriti, gli aiuti giusti alle piccole e medie imprese e alle famiglie per pagare i mutui saranno piccole briciole rispetto al macigno che blocca il mercato interbancario in Europa ed in Italia. E questo è compito dell'autorità della Banca centrale europea. E vengo alla terza e ultima riflessione, dando atto a tutti i Gruppi che hanno lavorato all'interno della Commissione finanze di serietà nel merito della discussione; atteggiamento che ci ha consentito di arrivare in Aula

Si è detto da più parti che occorre fare di più rispetto al decreto che venerdì scorso il Governo ha adottato per 5-6 miliardi, relativamente pochi, ma relativamente tanti perché concentrati sulle fasce più deboli. Ebbene, occorre tener presente un parametro di riferimento: chiunque voglia proporre seriamente

che ogni punto percentuale sui tassi d'interesse costa alla Repubblica italiana, ai cittadini italiani, 15 miliardi di euro in più di oneri finanziari sul debito pubblico. Ciò dimostra il velleitarismo e la demagogia

tuttavia, che la Presidenza è stata costretta a sospendere i lavori dell'Assemblea per venti minuti. La inviterei, pertanto, per il futuro, ad osservare una maggiore puntualità, in un rapporto di reciproco rispetto per il quale fin d'ora la ringrazio.

sulla prevenzione e cura dell'osteoporosi. Dopo l'illustrazione delle mozioni, ciascun Gruppo avrà a disposizione dieci minuti, comprensivi dei tempi della discussione e delle dichiarazioni di voto. Ha facoltà di parlare la senatrice Bianconi per illustrare la mozione n.

L'osteoporosi colpisce una donna su due dopo i 45 anni ed un uomo su cinque: sono dati estremamente allarmanti e ci fanno capire l'esatto confine di questa patologia. Le previsioni dell'Organizzazione mondiale della sanità sono molto preoccupanti poiché ci dicono che, entro cinquant'anni, in Italia potranno esserci circa 24 milioni di osteoporotici,

Purtroppo, anche in assenza di sintomi, la malattia avanza e l'osso diventa fragile fino a fratturarsi. Spesso è la frattura di una vertebra a permettere la prima diagnosi e quando ciò avviene la malattia è in stato avanzato e certamente la qualità della vita della persona cala drasticamente. Il Parlamento europeo ha mostrato un forte interessamento per questa patologia, sottolineando i danni sociali ed economici per chi ne è colpito. L'Europa, tra l'altro, considera l'Italia tra le aree a maggiore rischio osteoporotico, dando rilievo al quadro demografico caratterizzato da una vita media tra le più lunghe sia in Europa che nel mondo. Questa malattia comporta pesanti oneri finanziari: i costi delle spese socio-sanitarie ammontano a circa 2.600 miliardi di euro,

I soli costi ospedalieri delle fratture del femore, quindi solo di una parte dell'osso compromesso, si attestano ogni anno in Italia Purtroppo, non avendo dati certi, la fotografia della situazione non è precisa. Possiamo quindi avvicinarci per stime,

Nella XIV legislatura, la 12a Commissione permanente del Senato approvò, il 7 maggio 2003, il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva condotta dalla senatrice Boldi; documento analitico che, nelle sue indicazioni al Ministero della salute, chiedeva di inserire l'osteoporosi tra le malattie croniche e invalidanti e chiedeva di rivedere i criteri della Nota CUF n. 79 devo dire che molto si è fatto anche grazie al prezioso lavoro svolto dall'allora sottosegretario Cursi. Oggi, con questa mozione che speriamo venga approvata con voto unanime, desideriamo continuare sul solco tracciato, segnando anche dei passi significativi in avanti, riaccendendo soprattutto l'attenzione su questa patologia anche alla luce dei dati che ho esposto. A tale proposito, i proponenti della mozione richiedono in primo luogo la promozione di campagne informative sui corretti stili di vita. Infatti, appare fondamentale la prevenzione primaria, da attuarsi sin dall'infanzia, promuovendo stili di vita ed alimentari corretti, un'alimentazione ricca di calcio e di vitamina D, l'eliminazione dell'uso del tabacco - e noi sappiamo quanto questo rappresenti ancora una grande piaga

promuovere anche la cultura della prevenzione secondaria attraverso controlli specifici ed una corretta diagnosi precoce. In secondo luogo, si chiede di istituire il registro delle prime fratture. Questa è una una cosa estremamente semplice da fare perché al pronto soccorso ogni medico, nella sua scheda di dimissione, o quantomeno in cartella clinica, può evidenziare esattamente il tipo di patologia.

di individuare una specifica scheda di dimissione ospedaliera, la cosiddetta SDO, che permetta di vedere riconosciuti i propri diritti ad una giusta e corretta terapia. Signora Presidente, termino il mio intervento dichiarando fin da ora tutta la mia soddisfazione perché di queste tematiche si è lungamente parlato anche in Commissione sanità e, quindi, so che c'è unanime

ma quando si parla di salute e di prevenzione in modo particolare e concreto, volto a migliorare la qualità della vita delle persone, anche in quest'Aula diamo un grande segnale di unità al Paese. *(Generali

credo che sia doveroso un ringraziamento alla collega Bianconi che per prima ha avuto l'idea di presentare una mozione su questo argomento. Sostanzialmente concordo con quanto da lei esposto tant'è che noi della Lega Nord voteremo convintamente a favore della sua mozione. Desidero solamente rimarcare in questa nostra ulteriore mozione sullo stesso argomento alcuni punti particolarmente rilevanti, a partire dal fatto che l'osteoporosi costituisce un vero e proprio problema di salute pubblica, di regola associato a fratture da fragilità, che a loro volta si traducono in un elevato incremento della morbilità, in un vario grado di inabilità permanente e, nei casi più gravi, addirittura in un qualche eccesso di mortalità per le conseguenze stesse delle fratture patologiche. L'Italia è il Paese europeo con la più alta percentuale di popolazione anziana e, con l'aumento della durata della vita media, anche nel nostro Paese questa malattia sta assumendo una dimensione tutt'altro che trascurabile. Non esistono, inoltre, ad oggi dati certi sulla diffusione della patologia osteoporotica; ed emerge, infatti, una marcata discreparanza tra i riscontri epidemiologici degli studi clinici e le risultanze emerse dall'indagine multiscopo sulle famiglie del 2000 condotta dall'ISTAT. La discrepanza registrata può essere imputata anche alla natura spesso asintomatica della malattia dell'osteoporosi, che rende complessivamente poco attendibili i rilievi anamnestici. Il problema della scarsa consapevolezza della patologia osteoporotica è stato di recente evidenziato dallo studio pilota condotto nel 2003 nell'area di Firenze dall'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con la Regione Toscana e 1'ISTAT. Dallo studio, infatti, è emerso che solo una donna su due affetta da osteoporosi è a conoscenza della sua patologia; per gli uomini, la percentuale è addirittura di uno

non tanto ai costi diretti legati all'ospedalizzazione quanto ai costi indiretti dell'osteoporosi. L'indagine conoscitiva svolta dalla 12a Commissione permanente nella XIV legislatura

È tuttavia significativo osservare come le giornate di degenza per frattura del femore siano addirittura più numerose delle giornate di degenza per patologie sicuramente più importanti e nobili come l'infarto del miocardico e la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Rispettivamente l'osteoporosi determina circa il 25 per cento di ricoveri in più rispetto all'infarto miocardico e addirittura il 40 per cento in più rispetto alla BPCO. Molto più difficile appare la stima dei costi indiretti conseguenti alla patologia osteoporotica, derivanti dai giorni di assenza dal lavoro per malattia e quindi dalla mancata produttività, nonché dell'impatto della patologia sulla spesa privata per le prestazioni assistenziali non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale, come quelle legate alla riabilitazione, che molto frequentemente sono considerate extra LEA. Al fine di ridurre il costo sociale della patologia, un contributo determinante è dato dall'implementazione dell'attività di promozione alla salute basata sull'epidemiologia, sull'evidenza, sulle campagne di prevenzione e sull'opera di diagnosi precoce. I fattori genetici giustificano, infatti, circa il 70 per cento della variabilità individuale della massa ossea ad ogni età, per cui una spiccata familiarità per fratture osteoporotiche sicuramente giustifica uno *screening* precoce della malattia. L'osteoporosi e la frattura osteoporotica presentano, tuttavia, una patogenesi multifattoriale, in quanto, oltre ai fattori genetici, la propensione al rischio osteoporotico sembra essere determinata anche da fattori indipendenti, che sicuramente giustificano l'opportunità del ricorso a campagne informative e di sensibilizzazione ad ampio spettro su tutto il territorio nazionale. Per l'osteoporosi la prevenzione deve, infatti, cominciare in età precoce, in quanto è nell'adolescenza che l'apporto di calcio attraverso gli alimenti viene più efficacemente assorbito dall'organismo, contribuendo così al consolidarsi della massa ossea. È inoltre necessario che l'attività di prevenzione sia rivolta anche alle persone di sesso maschile, troppo spesso dimenticate, che mostrano a loro volta una più spiccata propensione a sottostimare il problema. Tutto ciò considerato, con la mozione presentata noi desidereremmo impegnare il Governo a promuovere un'implementazione degli studi epidemiologici relativi alla patologia osteoporotica al fine di rilevare l'incidenza di fratture o di determinare la prevalenza della malattia, nel caso promuovendo la stipula di un accordo presso la Conferenza permanente per i rapporti finalizzato a definire comuni obiettivi epidemiologici anche attraverso l'utilizzo dello strumento dei registri di patologia; a promuovere uno studio nazionale sui costi diretti (ospedalizzazione ed altre forme di assistenza a carico del Servizio sanitario nazionale), sui costi indiretti (legati, in particolare, alla morbilità), nonché sui costi privati sostenuti autonomamente dai cittadini per le spese per le prestazioni extra LEA. impegni a monitorare l'offerta assistenziale extraospedaliera presente nelle diverse Regioni in relazione all'osteoporosi, a promuovere l'adozione di specifici progetti di prevenzione sanitaria volti a diffondere l'assunzione di calcio e colecalciferolo (la cui assenza costituisce la principale causa della patologia osteoporotica) e a promuovere la diagnosi tempestiva della patologia attraverso la diffusione il più vasta possibile e con una tempistica reale, non sempre compatibile con i tempi d'attesa delle nostre strutture sanitarie - della densitometria ossea e dell'indagine mineralometrica (MOC), che consentono di misurare con precisione la densità del tessuto osseo. Infine, vorremmo porre l'accento sulla opportunità di promuovere campagne di sensibilizzazione specificamente rivolte a prevenire i rischi di una diffusione dell'osteoporosi tra le persone di sesso maschile.

e verranno proseguite. In merito poi al Registro delle fratture di fragilità e alla richiesta di una specifica scheda di dimissione ospedaliera, poiché

mi limito a dire che il Gruppo dell'Italia dei Valori è rimasto persuaso della bontà dell'iniziativa della senatrice Bianconi, approva la mozione e la voterà.

Signora Presidente, annuncio subito che il nostro voto sulla mozione

quelle avanzate nella prima. Reputo molto significativo, soprattutto per i tanti malati che soffrono di questa patologia, che nell'Aula del Senato si discuta dell'incidenza ed anche delle conseguenze che l'osteoporosi porta nella vita delle persone e nella nostra società. È un atto di attenzione, ma è anche un pressante invito che viene rivolto al Governo e alle Regioni a mettere in atto gli strumenti che sono necessari per ridurre l'incidenza di questa malattia, un'incidenza crescente, perché sappiamo che questa patologia è legata all'invecchiamento della popolazione ed in particolare al fattore di genere. Purtroppo, è recente la notizia - cui accennava anche il senatore Rizzi - che anche i giovani cominciano ad essere a rischio e a tale proposito vorrei citare i dati di un convegno promosso a Perugia dalla Società italiana dell'osteoporosi, del metabolismo

che c'è stato un indebolimento progressivo dello scheletro dei nostri ragazzi. Le ragioni di questo fatto sono da ricercarsi nella cattiva alimentazione e nella mancanza di movimento. Bisogna pertanto mettere in campo, a partire dalle scuole, iniziative che informino i ragazzi, orientandoli verso una corretta alimentazione e incentivandoli allo sport e al gioco con i coetanei. In caso contrario, il rischio è che questi giovani arrivino a trent'anni con un deficit del 15 per cento della massa ossea e a sessant'anni siano dei potenziali malati di osteoporosi.

che parta anche dalla formazione dei medici di medicina generale, che più di altri possono sensibilizzare i loro pazienti. È risaputo che l'osteoporosi è una malattia a forte incidenza di genere. Sono le donne le più colpite, per alcune ragioni che

Questi fattori portano a determinare una diversa incidenza delle complicanze, ovvero di fratture ossee nei due sessi. Si calcola infatti che il 40 per cento delle donne, a fronte del 12 per cento degli uomini, sopra i 50 anni avrà nei restanti anni di vita una frattura per fragilità ossea. Nelle strategie d'intervento occorre perciò una particolare attenzione alla questione di genere. nel documento: «Guadagnare salute», che definisce le strategie europee per la prevenzione e il controllo delle malattie croniche, si argomenta a lungo sull'incidenza di genere nello sviluppo e sull'andamento dei fattori di malattia. Nel nostro Paese purtroppo lo studio di questi fattori e anche di modelli di cura «al femminile» è ancora poco considerato, anche se le donne nel nostro Paese in questi 50 anni hanno fatto dei passi da gigante per quanto riguarda il loro inserimento nella società e nel mondo del lavoro, assumendo anche posizioni di responsabilità. Questo ha portato a molti cambiamenti negli stili di vita, alcuni dei quali influiscono negativamente sulla loro salute. Dipartimento per il genere e la salute della donna, nei documenti pubblicati sul tema mette in evidenza la sostanziale sottovalutazione della diversità femminile riguardo la salute e la diversità rispetto agli uomini dell'esposizione ai rischi sanitari. di sensibilizzazione richiesta nella mozione n. 5 al Governo non può prescindere dal fatto che le più colpite sono le donne e che in loro la malattia insorge in una età ancora giovane. L'osteoporosi è anche una malattia della vecchiaia. Preoccupa che nel Libro verde del ministro Sacconi si sottolinei come l'invecchiamento sempre più accentuato della nostra popolazione, con il conseguente aumento della non autosufficienza, sia uno dei fattori che fanno presumere il raddoppio, entro il 2050, della spesa sanitaria. D'altra parte, non possiamo non fare i conti con questo fattore di invecchiamento che il Presidente del Consiglio, onorevole Berlusconi, nella rivista scientifica della Fondazione San Raffaele ampiamente ripresa dalla stampa quotidiana), ha previsto possa farci arrivare addirittura a 120 anni nel giro di poco tempo. Ritengo che questo allungamento della vita non debba essere alla portata solo di chi sarà nelle condizioni economiche di curarsi, ma di tutti. Da qui la necessità di attuare e rafforzare i piani di prevenzione della non autosufficienza, proprio riducendo l'incidenza delle malattie croniche e invalidanti, tra cui l'osteoporosi. aveva inserito tra le aree prioritarie di intervento le malattie dell'invecchiamento e le malattie a morbilità elevata per le quali esistono prospettive di prevenzione, trattamento o ritardo

Quello che mi sento di chiedere è che tutto questo lavoro oggi non vada disperso, anche se reputo importanti gli obiettivi contenuti nelle mozioni, che sono stati qui raccolti dal Sottosegretario. Ben venga il Registro delle fratture di fragilità, perché è lo strumento per registrare quel tipo di fratture fratture derivanti dall'osteoporosi, piuttosto che da traumi. Ben venga anche l'istituzione di una scheda specifica per le dimissioni ospedaliere (SDO) per rassicurarci del fatto che questo poi comporti un automatico riconoscimento dei diritti di terapia. Mi auguro che il Ministro vorrà quanto prima convocare la Conferenza Stato-Regioni per chiedere loro impegno e definire dei piani in prospettiva. Curarsi oggi non è alla portata di tutti. Vi sono differenze fra Regione e Regione; spesso le medicine vengono date gratuitamente solo quando la malattia è molto avanzata. Se è vero come è vero che l'osteoporosi è una malattia cronica e i farmaci vanni assunti per molti anni, c'è anche un problema che riguarda la tollerabilità e la sicurezza dei pazienti che andrebbe verificata; inoltre, c'è un problema di costi. Consideriamo questa mozione, che impegna il Governo a darsi alcuni obiettivi per affrontare la questione osteoporosi, come un passo avanti utile e necessario. che con le Regioni vengano fatti gli accordi necessari perché queste iniziative possano essere attuate in tutto il Paese. Infine, è importante che i livelli essenziali di assistenza in via di revisione non smentiscano queste strategie e che ci sia un ampliamento degli effetti di questa iniziativa attraverso un potenziamento dell'azione di prevenzione, che va attuata attraverso piani e risorse adeguate. Il nostro voto - ripeto - sarà favorevole.

Piano sanitario nazionale aveva inserito tra le aree prioritarie di intervento le malattie dell'invecchiamento e le malattie a morbilità elevata per le quali esistono prospettive di prevenzione, trattamento o ritardo della comparsa (sostanzialmente l'osteoporosi e l'osteoartrosi).

il doppio ne sono previsti per il 2020 e ogni anno almeno 80.000 persone incorrono in una frattura di femore. Vi è l'esigenza di intervenire in maniera

dimostra ancora una volta, seppure ve ne fosse bisogno, la sensibilità a queste tematiche, ma soprattutto la dimostra in un percorso che sarà sicuramente irto di difficoltà, quale quello della verifica in sede di Conferenza Stato-Regioni dei due strumenti ricordati, che possono

di attuare sistematiche attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria tramite interventi in grado di affrontare la molteplicità di fattori che concorrono a determinare l'insorgenza di tale patologia: mantenere uno stile di vita sano con adeguata esposizione alla luce solare; evitare l'ingestione di alcolici e l'abitudine al fumo; aumentare l'introito di calcio con la dieta; mantenere un adeguato peso corporeo. È inoltre basilare il rafforzamento delle reti assistenziali. Occorre intervenire sulle Regioni per fare in modo che tali reti vengano rafforzate, non solo per i servizi che riescono a fornire, ma anche in termini numerici: sono ancora poche a livello di territorio. Si parla tanto di assistenza sul territorio, si dice sempre "meno "meno ospedali più territorio": questo è un caso in cui il territorio può e deve rispondere. Quindi, occorre una forte integrazione dei servizi sociali e sanitari per prevenire e migliorare le condizioni di disabilità che tale patologia

Signora Presidente, il 24 luglio di quest'anno, la Presidenza del Senato ha accolto un ordine del giorno, che ho presentato insieme ad alcuni colleghi, in particolare senatori radicali, che radicali, che vincolava la Presidenza stessa a pubblicare *on line* le dichiarazioni presentate dai senatori in riferimento ai propri redditi e alle proprie proprietà mobiliari e immobiliari. La ragione di questa iniziativa è evidente. La pubblicità prevista dalla legge del 1982 non è più adeguata rispetto a ciò che si intende oggi per pubblicità. Oggi la vera pubblicità è data dalla pubblicazione *on line*. quattro mesi di distanza, questo impegno assunto dalla Presidenza del Senato non è stato ancora onorato. Ho chiesto il motivo agli Uffici competenti e mi hanno risposto che la legge del 1982 prevede che la pubblicazione avvenga congiuntamente per le dichiarazioni dei senatori e per quelle dei deputati. Questa risposta però non mi sembra congrua, dal momento che l'adempimento dell'obbligo previsto dalla legge del 1982, nelle forme stabilite da quella norma, non impedisce affatto che la Presidenza del Senato, essendosi assunta l'impegno di fare qualcosa di più su questo terreno,

e magari prevedendo un meccanismo che consenta la tracciabilità di coloro che intendono accedere a questi dati. Chiedo che la Presidenza del Senato

Non si vede per quale motivo quella trasparenza debba valere per gli altri e non per noi. Senatore Ichino, la Presidenza ha presente l'ordine del giorno da lei richiamato. A tale riguardo, la informo che si stanno valutando le possibili soluzioni, sul piano normativo, all'esigenza da lei posta con le necessarie intese con l'altro ramo del Parlamento.

La seduta è tolta